convertito nella legge n. 133 del 2008) prevede per gli enti locali, quale sanzione per il mancato rispetto del Patto di stabilità nell'esercizio precedente, il divieto generalizzato di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Tale sanzione si applica dall'entrata in vigore del citato decreto-legge e, pertanto, la sua operatività non può risalire all'anno 2006. Di conseguenza, l'assunzione di personale (avvenuta nell'agosto con l'interrogazione non appare illegittima, sempre che il Comune in questione abbia effettivamente rispettato il patto di stabilità nel 2007. Aggiungo che, in ogni caso, l'assunzione deve essere compatibile con la specifica disciplina normativa prevista dall'articolo 1,

Pertanto, l'assunzione sarà legittima solo se inquadrata in un contesto più ampio, nel quale l'ente riesca ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità nell'esercizio in corso e la diminuzione del volume complessivo delle spese di personale rispetto a quelle sostenute nel 2007. Aggiungo, infine, che risulta che il Comune di Inzago abbia rispettato il Patto di stabilità interno sia nel 2007 che nel 2008.

le limitazioni imposte dall'ordinamento nazionale nei confronti di coloro i quali circolano in luoghi pubblici con il volto celato, come noto, sono dettate dall'articolo 85 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che sancisce il divieto di comparire mascherati, e dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, che, all'articolo 5, prescrive il divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo. In sede di interpretazione di tale normativa, l'assimilabilità delle due ipotesi (velature islamiche e travisamento in luogo pubblico) è stata sovente ritenuta controversa, soprattutto per ciò che concerne la possibilità di far rientrare nel divieto di travisamento la fattispecie della copertura del volto mediante il *burqa* o altra copertura similare, non potendosi parificare quest'ultimo ad una maschera, né ad un qualsiasi travestimento diretto volontariamente ad alterare i tratti somatici della persona. Ciò non toglie, peraltro, che anche nei confronti di coloro che indossano il *burqa*, o qualunque altra velatura, operano le limitazioni imposte dall'ordinamento a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, fra le quali rientrano gli obblighi di consentire e non ostacolare il riconoscimento della persona da parte degli agenti a ciò abilitati. Quest'ultima questione, in particolare, è venuta in evidenza in relazione all'applicazione del citato articolo 5 della legge n. 152 del 1975 che, come detto, vieta di prendere parte a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto. Rispetto a tale norma, la più recente legge 31 luglio 2005, n. 155, ha comportato solo un inasprimento di pena, senza tuttavia intervenire sul profilo contenutistico della disposizione. Preciso in proposito che, trattandosi di norma penale, ogni valutazione in merito all'ambito di operatività della stessa - come anche l'eventuale apprezzamento di particolari esimenti religiose - non può che appartenere all'esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria. Sottolineo, peraltro, che resta ovviamente ferma ed impregiudicata la facoltà delle Forze di polizia di attivare i propri poteri di identificazione, anche nei confronti della persona che circoli in luogo pubblico col volto coperto da un segno di fede religiosa, qualora esistano circostanze ambientali tali da costituire giustificato motivo di allarme per la sicurezza. In tal senso sono orientate le indicazioni e le direttive diramate sull'argomento dal Ministero dell'interno. Venendo ora allo specifico episodio citato dall'interrogante, riferisco che il 4 agosto scorso, con volo proveniente da New Delhi, sono giunte all'aeroporto di Malpensa, in transito verso Parigi, due donne che indossavano il *burqa*. Secondo le ordinarie procedure, le donne sono state sottoposte a quattro diversi controlli - tre specifici, attuati attraverso postazioni fisse ed uno in forma mobile - dai quali non sono emersi rilievi di sorta. In particolare, il primo controllo è avvenuto tra la zona di arrivo e la zona di transito dello scalo, dove, secondo quanto previsto dal Programma nazionale di sicurezza, vengono effettuate le ispezioni radioscopiche dei bagagli a mano, i passaggi sotto i portali e quant'altro è necessario per impedire l'ingresso sul territorio nazionale di armi, munizioni, esplosivi ed ogni ulteriore dispositivo che possa arrecare danno alla sicurezza. Superate queste verifiche, le due donne sono state sottoposte al controllo dei passaporti, coerentemente alle disposizioni interne (decreto legislativo n. 286 del 1998) ed europee (codice frontiere Schengen del 15 marzo 2006) che prevedono, tra l'altro, l'identificazione, l'accertamento dello scopo del viaggio e dei mezzi finanziari, il controllo presso le banche dati. Nello specifico, al momento dell'identificazione, a seguito dell'invito degli operatori a sollevare il velo sul volto, le donne non hanno opposto alcuna resistenza, per cui è stato possibile proseguire negli accertamenti, senza incontrare difficoltà di sorta. Le stesse, che viaggiavano con i rispettivi consorti, sono state quindi ammesse ai cancelli d'imbarco, in attesa del completamento delle operazioni per la prosecuzione del viaggio. Al momento dell'ingresso sull'aereo, sempre secondo le procedure del Programma nazionale di sicurezza, alle due passeggere veniva nuovamente richiesto di sollevare il velo, ai fini dell'identificazione e per il riscontro tra la carta di imbarco e il documento di identificazione. Anche quest'operazione, come già detto, è avvenuta senza alcun problema. Agli atti sono conservate le generalità delle due donne. Come è evidente, i controlli pianificati si sono svolti con estrema cura e il transito delle due donne sul territorio nazionale non ha determinato alcun significativo problema sotto il profilo della sicurezza pubblica. Soggiungo, inoltre, che l'eventuale richiesta di rimozione del velo durante il periodo di temporanea permanenza presso lo scalo aeroportuale sarebbe stata inutile ed avrebbe potuto essere percepita come vessatoria. Occorre però evidenziare che, nel nostro ordinamento, la facoltà (non l'obbligo) di identificazione non è rimessa all'arbitrio dei singoli operatori, ma va esercitata nei casi in cui ciò appare necessario, alla luce del principio che un ordinamento democratico deve riuscire a coniugare il massimo di sicurezza collettiva con il minor sacrificio possibile per le libertà individuali. È, comunque, cautela necessaria procedere all'identificazione nei luoghi in cui la presenza di una persona che occulta le proprie sembianze - e ciò che può portare indosso - può costituire un obiettivo fattore di rischio, così come tali circostanze integrano un valido motivo per impedire alla stessa persona l'accesso in altri luoghi sensibili, soprattutto ove vi siano concentrazioni di persone e giustificati motivi di allarme. Concludendo, sottolineo che nel caso di specie sono state garantite le esigenze di sicurezza delle persone in transito nell'aeroporto di Malpensa, attraverso la puntuale ed attenta attività delle Forze dell'ordine, che hanno agito secondo procedure operative pianificate e nel rispetto della vigente normativa.

Sicuramente, da quanto lei ha puntualmente e diligentemente riferito, è stata messa in atto ogni misura atta a prevenire eventuali pericoli che potessero derivare dalla presenza di persone non identificabili immediatamente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 15 ottobre ultimo scorso personale della Polizia municipale di Oriago di Mira in provincia di Venezia denunciava alla locale stazione dei carabinieri che ignoti, mediante un pennarello di colore nero, avevano imbrattato con una scritta, insulti, simboli celtici e la sigla "SS" un monumento dedicato alla memoria dei caduti del Secondo conflitto mondiale, ubicato in località Borbiago di quel comune all'interno di un'area privata, recintata e attigua alla corsia dell'autostrada A4. L'episodio segnalato è tuttora oggetto di indagini da parte dell'Arma dei carabinieri, coordinate dall'autorità giudiziaria competente: allo stato appare riconducibile ad un mero atto vandalico - peraltro di estrema gravità - come sembrerebbe rilevarsi dal fatto che non siano stati profanati altri monumenti alla memoria dei caduti del Secondo conflitto mondiale. Circa le iniziative per prevenire tali deprecabili episodi, è doveroso rilevare l'obiettiva difficoltà di un'attività preventiva in grado di impedire in modo assoluto fatti come quelli segnalati nella presente interrogazione. Ciò sia alla luce dell'elevatissimo numero dei possibili obiettivi distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia in quanto si tratta di gesti che, seppure gravissimi, non richiedono particolari attività preparatorie e, conseguentemente, risultano più difficilmente rilevabili attraverso una preventiva attività di informazione. Tuttavia, pur nella difficoltà di prevenire in assoluto condotte illecite come quelle descritte nell'interrogazione, anche per la loro estemporaneità, nondimeno lo sforzo delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine è comunque quello di predisporre ogni misura volta per volta diretta ad assicurare un capillare controllo del territorio e ad intensificare i servizi di informazione per il monitoraggio costante dell'attività dei gruppi politici più estremisti. Nello specifico, per tutti gli obiettivi sensibili che siano espressione di valori nazionali - quali quelli riconducibili alla lotta di Liberazione - già normalmente inclusi tra quelli da vigilare nel corso dei servizi di controllo del territorio, è stato disposto, a seguito di diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Venezia, un ulteriore potenziamento dell'attività di prevenzione generale, sensibilizzando a tal fine il personale operante. in concomitanza con la campagna elettorale appena conclusasi, sono state impartite direttive mirate, anche in conformità alle indicazioni ministeriali, per l'attuazione di una più diffusa e capillare attività di controllo del territorio per la quale sono stati richiesti e ottenuti specifici rinforzi.

persone portatrici di una cultura ben precisa, quella della vigliaccheria, che porta a nascondersi dietro l'anonimato, e noi sappiamo che questa è la cultura fascista: colpire rimanendo nell'ombra.

perché quotidianamente i muri sono imbrattati e si trovano in giro per le strade croci celtiche e tutta una serie di simboli

e la preoccupazione per molte intimidazioni a livello personale che circolano tra i ragazzi nelle scuole, soprattutto le medie superiori: il tasso di violenza sta crescendo e queste ne sono le manifestazioni esteriori. Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatta della risposta del Sottosegretario, perché essa vedo la riproposizione puntuale di indicazioni che alle forze dell'ordine vengono date in maniera precisa. Credo però vi sia bisogno di fare

le proprie opinioni, senza dover temere che qualcuno, in maniera vigliacca e nell'ombra, possa assumere nei suoi confronti atteggiamenti di ritorsione. Inviterei quindi il Governo a fare qualcosa di più incisivo,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 9 gennaio 2009, sono state introdotte rilevanti innovazioni alla normativa che regola le procedure di valutazione comparativa

ha previsto l'emanazione di un decreto per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici. Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto si afferma nell'interrogazione, il Governo non ha in alcun modo inteso bloccare le procedure in parola; infatti, dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha emanato, il 27 marzo 2009, il citato decreto, che è stato inoltrato a tutti gli atenei e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (Serie generale n. 84, del 10 aprile 2009). Pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'Avvocatura medesima, sono rimasti da chiarire alcuni aspetti critici in ordine allo svolgimento della complessa procedura da adottare; pertanto, al fine di evitare la formazione di contenzioso, è stata ravvisata l'opportunità di richiedere un secondo parere all'Avvocatura, reso il 16 luglio scorso. Il Ministero, sulla base dei pareri acquisiti, si accinge, sentita la Conferenza dei rettori, ad emanare un'apposita ordinanza a tutti gli atenei con l'indicazione degli adempimenti e delle relative date, per consentire la formazione delle commissioni giudicatrici nel più breve tempo possibile.

di ricerca»), ha ritenuto di modificare anche le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori,

Avete individuato una procedura complicatissima, tipica appunto dell'Italietta, nella quale si sovrappongono meccanismi tra loro contrastanti, ottenendo il risultato che le commissioni esaminatrici non sono in grado, come lei ha affermato in quest'Aula, di decollare. Anzi, avete paura che il meccanismo che voi stessi avete creato possa suscitare una reazione

in beffa. Signor Sottosegretario, con l'università non si scherza. Il reclutamento è importantissimo e mentre l'Italietta si mostra in questo modo ridicolo, molti vanno via

sul nostro Paese. Allora, per qualche giorno, tutti a rincorrerci per fare le dichiarazioni più belle sulla necessità di far rientrare i ricercatori e di voltare pagina con le procedure di reclutamento nel nostro Paese. Sottosegretario, così non va bene. Lo dica al suo Ministro; la informi che il Parlamento se ne accorge: non siamo tutti ingenui e stupidi; facciamo emergere queste gravissime contraddizioni. Nel frattempo, è necessario informare il nostro Paese di quello che accade. Anzi, noi dell'opposizione, da questo punto di vista, dovremmo fare molto di più, perché sul futuro dell'università e sul reclutamento ci giochiamo molta della nostra serietà e credibilità. Oggi tutto è bloccato; oggi chi aveva fatto domanda prima del vostro decreto non ha nessuna possibilità di essere valutato, di essere esaminato, di avere, nel proprio Paese, l'occasione per dimostrare se è adatto o no ad inserirsi nel circuito della selezione e, quindi, dell'università. È un fatto grave. Ne prenda atto. Informi il suo Ministro; le dica che in Parlamento ce ne siamo accorti, lo denunciamo, lo diremo in tutte le università italiane e faremo valere le buone ragioni di una università moderna,

faccio presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 636, ha previsto che il Ministro definisca annualmente criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e che i contributi siano erogati, in via prioritaria, alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro. Con il decreto ministeriale del 21 maggio 2007, che ha fissato nuovi criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007-2008 si è data attuazione alla predetta norma, stabilendo che gli importi da assegnare alle singole scuole venissero calcolati sulla base dei dati inseriti dalle stesse scuole paritarie in una apposita anagrafe nazionale, istituita per individuare le scuole dell'infanzia senza fini di lucro. II predetto decreto, relativamente alle scuole dell'infanzia, ha previsto che il 20 per cento della somma definita a livello nazionale fosse assegnata a tutte le scuole paritarie e l'80 per cento alle sezioni delle scuole paritarie senza fini di lucro. Si deve precisare che fino all'anno 2007 i capitoli di bilancio degli uffici scolastici regionali erano incrementati da risorse aggiuntive assegnate dal Ministero tramite la ripartizione di un fondo nazionale. Dall'anno 2008 detto fondo non è stato più previsto e le somme, con decreto del 28 dicembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio 2008, sono state direttamente e totalmente assegnate agli uffici scolastici regionali a copertura di tutto l'esercizio finanziario 2008 sulla base della spesa storica e non si è potuto tener conto dell'effettivo fabbisogno di ciascuna regione. Infatti, il dato determinante ai fini dei conteggi, vale a dire la qualificazione della scuola come scuola a fini di lucro o senza, non era assolutamente conosciuto dall'Amministrazione e pertanto è stato possibile quantificare il fabbisogno dopo le operazioni di inserimento dei dati nella sopraindicata anagrafe, conclusesi tra la fine di dicembre del 2007 e i primi mesi del 2008. I predetti uffici scolastici hanno utilizzato per l'anno scolastico 2007-2008 le somme assegnate nel bilancio 2007 (per quattro dodicesimi) e nel bilancio 2008 (per otto dodicesimi) provvedendo ad erogare i contributi sulla base dei conteggi effettuati dal sistema informatico che gestisce l'anagrafe nazionale. Dai dati inseriti nella predetta anagrafe si evince una forte prevalenza di scuole senza fini di lucro nell'Italia settentrionale e centro-settentrionale e una presenza di scuole senza fini di lucro nettamente inferiore nell'Italia meridionale. Questa situazione ha comportato la necessità per l'Amministrazione di effettuare, nell'anno 2009, le compensazioni tra Regioni, riducendo, di conseguenza, gli stanziamenti assegnati ad alcuni uffici scolastici regionali ed incrementandone altri. Peraltro, occorre tener presente che parte della riduzione degli stanziamenti assegnati agli uffici regionali nel 2009 è dovuta all'applicazione del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Premesso quanto sopra, per quanto concerne la situazione rappresentata dall'interrogante si deve precisare che per il corrente anno 2009, come è noto, è stato previsto uno stanziamento aggiuntivo di 120 milioni di euro a favore delle scuole paritarie. Detta somma è stata ripartita, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con i Ministeri per i rapporti con le Regioni e dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2009. In particolare, per l'ufficio scolastico regionale della Calabria è stata disposta l'assegnazione di ulteriori 2.215.274

primario delle scuole paritarie dell'infanzia presenti in Calabria, che sono dotate di 760 sezioni e garantiscono 14.787 famiglie, peraltro in un territorio particolarmente complesso e delicato, dove sia la politica che la pubblica amministrazione non godono di grandi consensi. Al di là di tutti gli altri problemi, credo che questo in particolare sia sentito dalle famiglie calabresi. Non posso ritenermi soddisfatto, onorevole Sottosegretario. Ritengo che il Governo possa fare sicuramente di più e pertanto mi auguro che nella prossima finanziaria ci possa essere una maggiore attenzione verso le scuole paritarie dell'infanzia presenti in Calabria.

a seguito del maltempo che, nei mesi di novembre e dicembre 2008, ha colpito il territorio nazionale, è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, lo stato di emergenza. Successivamente, in data 16 gennaio 2009, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008». Con questa ordinanza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono stati nominati commissari delegati per il superamento dell'emergenza, con il compito di accertare i danni provocati dall'ondata di maltempo, di adottare tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite, nonché di porre in essere ogni utile attività per l'urgente avvio della messa in sicurezza delle aree colpite e per gli interventi di prevenzione. Lo stesso provvedimento ha previsto, da parte dei commissari, la quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione della popolazione colpita, per la ripresa delle attività produttive ed economiche e per il ripristino dei beni immobili danneggiati. Inoltre, l'articolo 1 ha disposto che ciascun commissario delegato, sul proprio ambito regionale, sentiti i Comuni e le Province interessati, predisponga un piano generale degli interventi indifferibili e urgenti finalizzati al ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica, alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua e alla messa in sicurezza del territorio. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della suddetta ordinanza n. 3734, il Presidente della Regione Basilicata, commissario delegato, è stato autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito. In relazione all'aspetto idrogeologico il territorio della Regione Basilicata rientra nelle zone di competenza delle Autorità di bacino interregionali della Basilicata, della Puglia, del del Fiume Lao e del Fiume Sele, le quali hanno approvato e adottato i rispettivi Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengono le perimetrazioni delle aree riconosciute a pericolosità e/o rischio da frana o da alluvione. Su dette aree sono vigenti norme di uso del territorio, in attesa, ove possibile, della mitigazione dei rischi idrogeologici attraverso le opere di difesa del suolo, secondo le priorità di intervento. Inoltre, la Regione Basilicata non ha ancora predisposto il Piano per la difesa delle coste con il quale, attraverso l'individuazione degli squilibri morfologici costieri e delle relative cause, si potranno stabilire, in maniera organica, tutte le azioni per l'uso e la difesa dall'erosione del territorio costiero. In Italia il problema dell'arretramento delle spiagge riveste particolare importanza e, in molti casi, gli equilibri morfologici lungo i litorali sono fortemente modificati, sia per il mancato apporto solido da parte dei fiumi che per l'interruzione del trasporto litoraneo di sabbie da parte di opere marittime. Questi fenomeni, spesso combinati, generano lungo i tratti costieri, nella rispettiva porzione sommersa, un *deficit* di volumi e di masse di sabbie di entità elevatissima, procurando, di conseguenza, una progressiva riduzione delle difese naturali. I tratti di spiagge italiane che risultano in arretramento sono circa 1.600 chilometri, di cui 20 chilometri interessano la Basilicata che, comunque, è tra le Regioni meno colpite dal fenomeno. Per quanto riguarda la difesa del suolo, i fondi messi a disposizione dalle leggi finanziarie su scala nazionale sono ogni anno molto esigui se confrontati con gli oltre 40 miliardi di euro del fabbisogno economico necessario per la sistemazione dei bacini idrografici e delle aree a rischio idrogeologico. Per la messa in sicurezza dei beni esposti a rischio di erosione costiera, le necessità economiche, in via preliminare, sono di oltre 4 miliardi di euro, mentre il fabbisogno complessivo, stimato nei PAI del 2006 per la sistemazione dei bacini idrografici della Regione Basilicata, è superiore a 3.000 milioni di euro. Nel 2005 sono stati resi disponibili ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasferite agli enti locali e alle Regioni, risorse economiche pari a 275 milioni di euro, dei quali circa 8,5 milioni sono stati attribuiti alla Regione Basilicata per la riduzione del rischio idrogeologico. Le disponibilità finanziarie degli anni 2006 e 2007 sono state, rispettivamente, di circa 222 e di 241 milioni di euro e, di questi, sono stati assegnati alla Regione Basilicata, per l'anno 2006, oltre 8,3 milioni di euro, mentre per l'anno 2007 circa 5,8 milioni di euro. Anche nel 2008 i finanziamenti disponibili sono stati di 252 milioni, mentre sono stati attribuiti alla predetta Regione circa 5,8 milioni di euro. Infine, si fa presente

Signor Presidente, ringrazio il gentile Sottosegretario per l'informativa resa,

sette mesi fa. Con tale interrogazione si chiedeva al Governo, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Basilicata nella prima decade di dicembre, quali iniziative, di concerto con la Regione stessa e con gli enti locali gli enti locali colpiti da tali eventi, intendeva intraprendere al fine di predisporre un piano di finanziamento straordinario per la messa in sicurezza degli immobili, e se non riteneva opportuno erogare un contributo a titolo di indennizzo in favore dei titolari delle attività agricole e delle altre attività produttive e commerciali, in particolare le attività turistiche. Sottosegretario, a questo quadro già molto negativo devono aggiungersi i danni provocati alle imprese agricole dalle ricorrenti calamità naturali e da altri imprevedibili eventi dannosi, non ultima la grandinata

è ancora in attesa del decreto ministeriale di riconoscimento dei danni da parte del Governo. Inevitabili, naturalmente, e pesanti sono stati i contraccolpi negativi sulla base produttiva; tra questi, per quanto riguarda il comparto agricolo, la riduzione delle polizze assicurative in contesti produttivi come quelli della Basilicata, già in sofferenza per problemi di Il fenomeno chiaramente è stato indotto dal mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, che è venuto purtroppo a coincidere con varie calamità naturali che si sono verificate, verificate, soprattutto negli ultimi mesi, trasversalmente su tutto il territorio nazionale, in un contesto in cui gli agricoltori, in molti casi, risultavano già parzialmente o totalmente scoperti dalle polizze assicurative. Altre motivazioni, signor Sottosegretario, della mia insoddisfazione alle risposte ricevute in Aula traggono origine da una serie di informazioni e di documenti assunti, durante tutti questi mesi, presso i competenti uffici

del dicembre 2008, provvedessero, tra l'altro, a quantificare le spese sostenute dalle amministrazioni per interventi urgenti effettuati entro la data del 23 gennaio così come stabiliva che altre misure e azioni dovessero essere assunte in favore dei soggetti privati danneggiati (ai quali, da questo punto di vista, non è stata data alcuna risposta da parte del Governo nazionale) e per interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Devo dire che soltanto in data 24 marzo è stata richiesta alle Regioni la prevista intesa su uno schema di ordinanza contenente un'ipotesi di riparto della somma stanziata, pari a 85 milioni di euro. La Regione Basilicata con nota in data 8 aprile 2009, ha rappresentato le proprie spese effettive secondo quanto disposto dall'ordinanza e poi, con successiva nota presidenziale del 16 aprile, la stessa Regione ha espresso invece parere negativo sull'intesa in quanto l'ipotesi di riparto, peraltro relativa solo alla misura prevista dalla lettera *a)*, la vedeva esclusa rispetto alle altre Regioni; con la stessa nota faceva rilevare che le somme somme ivi riportate erano solo presunte e indicative e quindi non rispondenti al dettato normativo, ma precisava anche di poter esprimere un'intesa favorevole nel caso fosse stata considerata la propria informativa sulle spese, peraltro

si è proceduto alla formale assegnazione di somme a tutte le Regioni tranne che alla Basilicata solo sulla base di comunicazioni forse più tempestive, signor Presidente, ma certamente non documentate né basate sulle previste certificazioni,

si chiede al Governo intanto di verificare se sono vere le informazioni recentemente assunte che dimostrerebbero la sussistenza di rilevanti economie derivanti dal notevole scarto tra le spese effettivamente documentate da alcune Regioni assegnatarie di fondi e quelle indicate inizialmente e, in caso affermativo, di procedere ad una rimodulazione delle somme disponibili, assegnando a tutte le Regioni risorse finanziarie nella misura corretta, secondo quanto disposto dall'OPCM n. Ciò anche in considerazione del fatto che la Regione Basilicata ha provveduto tempestivamente, con ordinanza del Presidente commissario delegato, emanata in febbraio, a finanziare interventi urgenti per il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate danneggiate e per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro. conclusione, a fronte dei gravi danni subiti da strutture e infrastrutture pubbliche e private in molti territori comunali della Basilicata, nel periodo che va da dicembre 2008 a gennaio 2009, e pur in presenza di un'ordinanza che ha dichiarato

vuole dare impulso al Governo nazionale e ovviamente, per la parte di competenza, che non è di poco momento, ai Governi territoriali (in questo caso la Regione Basilicata),

Nel cogliere l'occasione per dire che nel Mezzogiorno occorre mettere a sistema tutta la *governance* che in questi anni forse non sempre opportunamente ha governato questi schemi idrografici (su questo bisognerebbe fare una riflessione per capire quanto con l'avvento delle Regioni queste problematiche hanno avuto l'attenzione

una verifica stringente non solo sulla quantità delle risorse da mettere a disposizione, ma anche sulle modalità con cui le nuove autorità si stanno applicando per difendere il territorio, che è un bene prezioso per ogni ipotesi di sviluppo.

troppo facile continuare, anche se vedo che c'è un impegno del presidente Schifani e di tutti voi. Speriamo di risolvere questo problema,

e a Roma, dove è stato sequestrato un patrimonio immobiliare valutato in circa 200 milioni di euro. Sono state colpite cosche mafiose dei Bellocco e di altre famiglie che gravitano nel basso Lazio e, nel caso specifico,

e istituzioni. Il prefetto Frattasi ha denunciato da tempo questo fatto; i 17 arresti di due settimane fa tra politici locali e funzionari comunali non sono bastati a far sciogliere il Comune. Leggo con soddisfazione che il ministro Alfano dice che l'operazione della 'ndrangheta al «Café de Paris» de Paris» è «l'ennesima dimostrazione che la strategia individuata dal Governo, sul fronte della criminalità organizzata, è quella giusta». Faccio presente a lei, Presidente, e al Ministro che questa operazione è frutto delle intercettazioni telefoniche capillari che sono seguite per molti mesi e ricordo che questo Governo vuole impedire proprio queste intercettazioni, che speriamo non a settembre. Ecco, invito il ministro Alfano a riflettere su quanto da lui stesso detto: «questa operazione è l'ennesima dimostrazione che la strategia individuata dal Governo,» (oggi, ancora con il permesso delle intercettazioni) «sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, è quella giusta». Speriamo resti sempre giusta, non solo con riferimento alla criminalità, ma per tutto ciò che concerne all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che, guarda caso, portano sempre agli arresti eccellenti.